relativi allo svolgimento, da parte del sindaco di Catania, del mandato conferitogli di Commissario delegato per l'emergenza del traffico e del rischio sismico, facendo riferimento in particolare agli obiettivi della sua azione e ad alcuni aspetti di carattere gestionale, ivi inclusi quelli relativi alla rendicontazione, e riferendosi altresì ad alcuni interventi tra i quali, di particolare rilievo, quelli previsti per - diciamo così - la sistemazione urbanistica di una piazza catanese.

il Governo ritiene meritevoli di maggiore considerazione. Intendo richiamare a tal proposito che il succedersi dell'attribuzione al sindaco di Catania delle funzioni di Commissario delegato con diverse ordinanze della Protezione civile (la prima con riferimento ai poteri straordinari derogatori, l'altra, invece, del dicembre scorso, con riferimento all'attività in regime ordinario di completamento e di realizzazione delle opere nel frattempo programmate) ha avuto un'interruzione il 30 aprile di quest'anno (successivamente dunque alla data di presentazione dell'interrogazione) perché il Presidente del Consiglio dei ministri non ha prorogato

Questa circostanza non è secondaria ai fini di alcuni dei quesiti rivolti dagli onorevoli interroganti, il primo dei quali quello sul quale ritengo di dovermi soffermare ulteriormente - si riferisce alle attività che sono state predisposte per il parcheggio di piazza Europa.

perché il Commissario delegato si è avvalso della procedura del *project financing* con la quale, al correlato vantaggio per la pubblica amministrazione di non dover provvedere all'onere finanziario di una determinata opera, deve tuttavia corrispondere un vantaggio economico per i finanziatori. Da questa formula scelta dal Commissario delegato sono scaturiti una serie di effetti legati sia alla alla costituzione dell'associazione temporanea di impresa che si è candidata a sostenere gli oneri per la realizzazione del parcheggio, sia alle modalità di gestione e di scelta delle opere relative: se cioè dovessero essere interrate o se nella parte sopravveniente ci dovessero essere altri manufatti (centro commerciale o altro). In proposito sono state fatte diverse ipotesi. In realtà, la soluzione adottata dal Commissario delegato appare di dubbia legittimità,

degli stalli realizzati, distribuiti su due livelli sotterranei. Non è stata ritenuta percorribile l'opzione di realizzare superfici commerciali all'interno della struttura, Le superfici commerciali, d'altra parte, non potevano essere realizzate in superficie, perché nel bando del *project* *financing* non era prevista alcuna realizzabilità di superfici sovrastanti, ma ci si limitava alla ipotesi di realizzazione di parcheggi totalmente interrati. A questo punto, pur ponendosi evidenti questioni di traffico, non si riuscirebbe a comprendere appieno la connessione tra l'emergenza traffico e la realizzazione del centro commerciale in sostituzione di aree adibite a parcheggio, perché questa sembrerebbe rispondere ad un'altra finalità. Peraltro, gli uffici del Dipartimento della protezione civile hanno sottolineato che sussistono dubbi di legittimità relativi alle procedure firmate dal responsabile unico del procedimento;

del Dipartimento della protezione civile, non poteva essere subdelegata ad altro funzionario o responsabile della pubblica amministrazione. L'associazione temporanea di impresa ha inoltre mutato in corso di gara la sua composizione. Sulla materia, segnalata più volte con un carteggio anche dal prefetto di Catania (che ha sollevato la dubbia legittimità delle procedure adottate dal

in relazione alle richiamate scadenze relative alla sovrapposizione delle funzioni di sindaco e di commissario delegato. In riscontro alle citate osservazioni, il sindaco di Catania, con nota del 24 agosto, ha comunicato di avere investito l'avvocatura comunale, riservandosi di comunicare le ulteriori determinazioni al Dipartimento.

risorse finanziarie erogate non dalla Protezione civile, ma da altri enti. Le funzioni di commissario erano relative soltanto alla possibilità di gestire in deroga gli interventi. Però non c'è dubbio che, così come per gli altri commissari che si occupano di vicende analoghe, bisogna riportare ad una qualche sede di controllo contabile l'utilizzazione delle risorse; il Dipartimento della protezione civile chiederà pertanto generale dello Stato di utilizzare degli strumenti di accertamento dell'uso e della destinazione delle risorse in materia. ultimo aspetto: alla conclusione delle indagini della magistratura, soprattutto di quella contabile, la Presidenza si riserva di affidare l'eventuale gestione stralcio delle iniziative in corso di completamento ad un soggetto un soggetto qualificato, per provvedere agli adempimenti di conseguenza. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, la collega Anna Finocchiaro ed io esprimiamo apprezzamento e soddisfazione per la risposta fornita dal Governo alla nostra interrogazione. Non siamo affatto contrari, in linea di principio, all'uso eccezionale della dichiarazione dello stato di emergenza e all'intervento di protezione civile per opere che abbiano una natura preventiva, effettivamente preventiva, allo scopo di ridurre i danni di un eventuale evento sismico di particolare gravità in una zona ad alto rischio come quella della nostra città. Sappiamo che questo, però, è un evento assolutamente eccezionale dell'ordinamento e che non si può utilizzare lo strumento della Protezione civile per opere che non abbiano l'esclusiva connotazione di interventi tendenti a ridurre il danno sismico. La ragione per la quale avevamo presentato questa interrogazione era esattamente quella di segnalare al Governo che nei quattro anni in cui il Commissario straordinario e il responsabile dell'ufficio hanno operato a Catania, sulla base dell'ordinanza di Protezione civile, in realtà si è svolta una serie di interventi che con il rischio sismico avevano poco o pochissimo a che vedere. Le nostre preoccupazioni sono state puntualmente esposte e riteniamo che avevamo ragione, tant'è vero che nei giorni scorsi la magistratura penale è intervenuta ponendo sotto sequestro, in particolare, due dei in particolare, due dei cantieri che erano stati aperti nonostante l'opposizione al Consiglio comunale nella città avesse più volte segnalato l'irregolarità, nonostante l'irregolarità fosse stata evidenziata nell'interrogazione della collega Finocchiaro e mia, nonostante (voglio sottolinearlo) l'irregolarità e l'illegittimità fossero state rilevate anche da autorevoli organismi, a partire dal collegio di difesa dello stesso Comune, dalla prefettura di Catania e dal Commissario per la protezione civile. Naturalmente la vicenda adesso farà il suo corso sotto il profilo dell'indagine. Certo, ci dispiace che la città oggi paghi un prezzo salatissimo per un cantiere aperto in una delle zone più importanti, che resterà in questa condizione, e che il prezzo sarà pagato dai cittadini.

che tutti gli interventi siano stati fatti, sostanzialmente, senza discutere, prescindendo dalle implicazioni urbanistiche dei lavori pubblici e, naturalmente, in termini del piano commerciale della città. È impensabile immaginare di fare interventi che vengono spacciati come opere di protezione civile per poi realizzare centri commerciali in zone ad altissimo pregio: questo è francamente inaccettabile. Riteniamo, allora, molto importante quanto ci dice oggi il Governo circa la confermata illegittimità di questo tipo di interventi.

Ci fa piacere l'impegno che viene assunto, cioè che sarà la Ragioneria dello Stato a chiedere tutti questi elementi, poiché nessuno - né la Protezione civile a livello nazionale, né il Consiglio comunale della città - era stato informato di come queste risorse fossero state utilizzate. Infine, troviamo assolutamente necessario che, completato l'*iter* degli interventi della magistratura, come ha detto il Sottosegretario, possa essere nominato un

ringrazio per la sua costante attenzione alle problematiche legate al patrimonio culturale del territorio toscano in generale, e fiorentino nello specifico.

del bilancio, una serie di spese per potenziare le misure di sicurezza nel Museo del Bargello, tra cui l'installazione di un *metal detector* all'ingresso e l'adeguamento del corpo di guardia. Inoltre, le vetrine della sala interessata dall'ultimo furto sono state dotate di un allarme volumetrico più sofisticato

dei Silvestrini del Museo di San Marco saranno rafforzati gli impianti di sicurezza che andranno ad aggiungersi al sistema TVCC. Sono inoltre in programma ed in alcuni casi già in fase di attuazione interventi atti ad aggiornare ed incrementare i sistemi di sicurezza dei musei del Polo museale fiorentino, finanziati nell'ambito della programmazione ordinaria 2007. Per quanto concerne più in generale l'aspetto della conservazione del patrimonio artistico fiorentino, in linea con quanto previsto dalle priorità stabilite dal Ministro nella direttiva per l'anno 2007, si richiama l'obiettivo strategico del miglioramento del sistema di sicurezza dei musei, dei monumenti, e delle aree archeologiche per prevenire attività criminose e/o terroristiche. In coerenza con tale direttiva

garantire una idonea conservazione delle opere. Per rafforzare la tutela penale del patrimonio culturale anche attraverso la rivisitazione delle sanzioni penali contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, il Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 ha approvato, su proposta del ministro Rutelli, il disegno di legge di delega al Governo per la riforma delle sanzioni penali in materia di reati contro il patrimonio culturale e del paesaggio. Le innovazioni proposte in materia di beni culturali consistono in specifiche aggravanti per il reato di danneggiamento e di furto d'arte quando abbiano ad oggetto beni culturali nell'inasprimento delle pene per la ricerca archeologica abusiva, nell'estensione del reato di ricettazione a chi detiene beni culturali di provenienza illecita, nell'aumento delle pene per il delitto di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale, nell'estensione del reato a chi detiene illecitamente il bene all'estero; nell'istituzione della fattispecie del riciclaggio in relazione ad operazioni sui beni culturali, nella previsione che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, a discrezione del giudice, al risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o ancora alla prestazione di attività socialmente utile non retribuita, nel rafforzamento infine dei poteri d'indagine per il perseguimento

costruito una sequenza di fatti che evidenziano un problema di sicurezza. Si tratta di una sequenza di furti e danneggiamenti, verificatisi il 6 giugno 2006, il 13 luglio 2006, il 22 luglio 2006, il 16 ottobre 2006

Ma c'è anche un'altra sequenza che potremmo scrivere, di questi giorni, che denuncia un problema di scarsa manutenzione.

se invece il Ministero è più orientato verso la promozione dell'immagine si creano dei problemi, anche perché l'unico intervento del ministro Rutelli è stato quello di venire a Firenze e portarci via per alcuni mesi l'«Annunciazione», creando altre preoccupazioni in termini di sicurezza. Intendo dire che da parte del Ministero per i beni culturali non una politica "gigiona" del prestito delle opere d'arte all'estero, ma un impegno costante, assiduo, centrato sulla tutela e la conservazione del patrimonio artistico. Signor Sottosegretario, prendo atto delle sue dichiarazioni e dei suoi impegni e la ringrazio nuovamente.

previdenza sociale*. In riferimento al quesito sollevato dal senatore Iovene, inerente la situazione logistica e strutturale della sede dell'INPS di Vibo Valentia, rendo note le informazioni ricevute dall'Istituto che, in via preliminare, ci dice che l'intera problematica è da tempo all'attenzione dei suoi uffici. sarebbe stato individuato uno stabile, di nuova costruzione, idoneo a ricevere gli uffici della sede INPS in argomento. L'Istituto ha però ribadito la necessità di un'approfondita valutazione in ordine ai costi che tale operazione richiederebbe, in considerazione dei tagli di natura finanziaria che ha subito. In particolare sono state previste, per le amministrazioni pubbliche, una serie di misure finalizzate al contenimento della spesa, anche attraverso la razionalizzazione delle strutture logistiche. Si fa comunque presente che la vicenda è seguita dai competenti uffici dell'Istituto, non soltanto a livello centrale ma anche a livello regionale e che vi è la volontà di mettere a punto tutte le procedure necessarie per pervenire, quanto prima, alla soluzione del problema prospettato, anche attraverso lo sviluppo di sinergie con altre amministrazioni. In riferimento invece all'interrogazione sul programma di sviluppo dell'area G.A.L. Serre Vibonesi s.r.l. di Serra San Bruno, l'articolo 1-*ter* della legge n. 236 del 1993 ha istituito presso il Ministero del lavoro un fondo apposito per lo sviluppo al fine di consentire la realizzazione, nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge, di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale. dei ministri n. 773 del 1993, sono stati dettati i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui trattasi, mentre con decreto del Ministro del lavoro del 31 maggio è stato approvato il programma finalizzato allo sviluppo economico dell'area della Comunità montana delle Serre Vibonesi, presentato dalla società G.A.L. Serre Vibonesi. Per la realizzazione del programma in argomento è stata stipulata, il 31 luglio 2000, una convenzione (cui è seguìto un protocollo aggiuntivo) tra il Ministero del lavoro e la società in parola. Tale atto disciplina, tra l'altro, anche le modalità di erogazione delle provvidenze ed i controlli da effettuare, prevedendo, in particolare, che il pagamento del saldo cento sia subordinato alla verifica amministrativo-contabile sulla rendicontazione delle spese, da effettuarsi da parte del reparto operativo del Comando dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro. va rilevato, come già evidenziato dal senatore Iovene nell'atto ispettivo in discussione, che nell'anno 2006 le attività di verifica sono risultate drasticamente ridotte a causa della contrazione delle risorse destinate destinate alle missioni degli ispettori. Sono in grado di informare che la situazione appare adesso sbloccata, in quanto le diverse direzioni regionali del lavoro, con decreto del Ministro del lavoro dello scorso 13 luglio, sono state incaricate di effettuare il rendiconto delle spese ai fini dell'erogazione del saldo dei programmi in argomento. In particolare, per quanto interessa in questa sede, la direzione regionale del lavoro di Reggio Calabria, competente relativamente alla società consortile G.A.L. Serre Vibonesi, il cui programma, come previsto dalla citata convenzione del 31 luglio 2000, si sarebbe dovuto concludere il 31 luglio 2006, si è già attivata per l'effettuazione dei controlli ed ha chiesto alla competente direzione generale del Ministero, la documentazione relativa alla suddetta convenzione. Sono stati chiesti, altresì, eventuali atti di verifiche effettuate dal reparto operativo del Comando dei carabinieri

gli interessi e gli oneri bancari dovuti all'indebitamento per la mancata erogazione dell'ultima quota di finanziamento si rischia - appunto - di vanificare il senso stesso dell'iniziativa.

lavorare nella tranquillità e nella serenità che sarebbero necessarie. Trattandosi di una realtà particolarmente delicata dal punto di vista economico ed occupazionale, questo richiede una maggiore attenzione. Ecco perché prendo atto che finalmente la situazione dopo molti mesi si è sbloccata, però chiedo che si faccia un ulteriore sforzo affinché effettivamente queste imprese ricevano le risposte che attendono da molto tempo e che meritano.